Signora Presidente, onorevoli senatori, il nostro Paese è caratterizzato da uno dei sistemi ambientali e paesaggistici di maggior pregio, ma risulta essere anche tra i più fragili e delicati. La pressione turistica e antropica che alcuni tratti di costa, soprattutto nelle isole minori, nelle aree marine protette e nelle aree marine di reperimento nei periodi estivi rischia di compromettere questo grande patrimonio di inestimabile valore. I flussi turistici non regolati rischiano, infatti, di aggredire il territorio

Si aggiunga, inoltre, che tali aree soffrono di una cronica carenza infrastrutturale, anche perché su molte isole minori e in vari tratti di costa sarebbe un delitto realizzare infrastrutture pesanti;

Il disegno di legge approvato dalla Commissione in sede referente mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane, delle aree marine protette e di reperimento e di particolari tratti di costa, che le doti di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. In questo modo si potrebbero dotare le coste italiane di posti barca in porticcioli *off shore* per l'attracco, e dotare queste realtà di servizi per la nautica da diporto che consentano una corretta fruizione del litorale e dell'entroterra. Un campo di ormeggio così delineato avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela del fondale marino. Il parco boe nasce infatti con la specifica finalità specifica finalità di limitare, se non eliminare del tutto, gli ancoraggi sulle praterie di posidonia oceanica o comunque in aree con fondali protetti. Durante la stagione estiva

Il problema degli ancoraggi è alla ribalta delle cronache scientifiche come uno dei principali fattori di impatto sull'ecosistema di posidonia; un fenomeno che diventa sempre più allarmante ed evidente, soprattutto - come ho già sottolineato - nella stagione estiva. Ricerche e studi effettuati hanno messo in evidenza la necessità di ovviare a tale problema per ridurne l'impatto ed esistono soluzioni di vario tipo per la realizzazione di campi boe, al momento l'unica alternativa accettabile al divieto assoluto di ancoraggio. La regolamentazione degli ancoraggi e degli accessi nelle aree protette, oltre a rispondere alla predetta esigenza ambientale, si rende necessaria per far fronte alla difficoltà degli approdi, particolarmente sentita nel periodo estivo.

Nell'illustrare i contenuti dell'articolato, si fa presente che l'approvazione di taluni emendamenti risponde alle indicazioni contenute nei pareri resi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente. In In particolare, l'articolo 1 prevede che, allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto nelle zone di riserva generale e parziale; tali progetti sono sottoposti al parere della locale capitaneria di porto. Vengono altresì delineate le finalità dei campi di ormeggio, ravvisate nella riduzione del fenomeno di aratura dei fondali, vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; nell'erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento nell'area, determinato dal numero di gavitelli disponibili, e nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio

della boa e non a quella degli ormeggiatori, come a volte accade. In tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedono alla definizione di tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e alla destinazione di una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni a propulsione velica; all'individuazione, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali stessi, ai fini di assicurare un minore impatto ambientale; all'adozione di adeguati sistemi, anche tecnologicamente avanzati (ad esempio le boe telematiche) per il monitoraggio remoto delle boe e dei pali a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento. inoltre prevista anche per i Comuni - è questa una novità importante - che non siano ricompresi nelle aree marine protette o di reperimento, la cui estensione territoriale ricada in tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, la facoltà di istituire campi di ormeggio attrezzati. In tal caso i Comuni dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché lo studio di incidenza nelle aree appartenenti alla rete «Natura 2000». L'articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento, all'interno delle quali i Comuni, in regime di esenzione concessoria e con la facoltà di affidare l'allestimento e la manutenzione a terzi, possono istituire i campi di ormeggio secondo i criteri e le finalità individuati dall'articolo 1. L'articolo 3, infine, stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i Comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.

Signor Presidente, onorevoli senatori, pochissimi provvedimenti ambientali e ancor meno disegni di legge di iniziativa parlamentare sono approdati in Aula dall'inizio di questa legislatura, caratterizzata da un predominio assoluto del Governo nella formulazione dei testi normativi da sottoporre al voto. Oltre due terzi delle leggi ordinarie sinora approvate, infatti, sono di origine governativa - compresi i decreti-legge e le ratifiche di trattati internazionali relegando al ruolo di spettatori i parlamentari appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione. È quindi un fatto da salutare positivamente la circostanza che la Commissione ambiente del Senato abbia licenziato un disegno di legge presentato dall'opposizione. Ci si augura che questo esempio spinga il Ministro dell'ambiente ad una maggiore attività e presenza legislativa sui temi di sua competenza, fra i quali rientra indubbiamente la tutela del mare. Nei giorni in cui l'importante ritrovamento del relitto affondato nelle acque calabresi a largo di Cetraro fa sperare a molti nella possibilità di affrontare con nuovo vigore le inchieste sulle cosiddette ecomafie e su una pratica - purtroppo assai diffusa che ha visto tra gli anni Ottanta e Novanta qualche decina di navi affondare nei punti più profondi del Mediterraneo, la tutela del mare è un elemento importante della salvaguardia ambientale più generale, coinvolgendo anche l'aspetto turistico ed economico della gestione del paesaggio e dei beni naturali del nostro Paese. Il nostro Paese, come il relatore ha rilevato, è caratterizzato da un sistema ambientale e paesaggistico di grande pregio quanto fragile e delicato. Gli episodi di questa estate, sui quali spetterà alla magistratura accertare le eventuali responsabilità penali, presentano come caratteristica comune un elemento preoccupante: la difficoltà, ancora forte ed anzi sempre più acuta, che sembrano incontrare le istituzioni nel presidio del territorio e, con tale presidio, nel contrasto preventivo alle attività illecite. Lo sversamento e l'abbandono di rifiuti lungo le coste, o addirittura direttamente nelle acque marine, si è rivelato attività ancora tanto frequente e redditizia quanto poco contrastata; e quando ciò avviene non è certo per una mancanza di norme. Se un intervento di tipo legislativo è necessario, esso consiste nell'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale, seguendo la proposta avanzata dal Governo Prodi nella scorsa legislatura. Quel che piuttosto viene seriamente messo a rischio dalla inesorabile contrazione delle risorse per il mare e dai tagli ripetuti ai trasferimenti verso le Regioni, gli enti locali e verso lo stesso Ministero dell'ambiente della legge finanziaria una contrazione di risorse assegnate del 18 per cento in un anno e, in termini reali, di quasi il 50 per cento in applicazione al decreto-legge n. 112 del 2008) è il livello pratico e operativo delle attività di prevenzione, repressione e monitoraggio previste dalla legge I problemi della flotta di unità specializzate antinquinamento del Ministero si sono posti questa estate in una fase molto acuta della fragilità dell'ecosistema marino, aggredito in Toscana, in Friuli, in Calabria, a Capri, a Ischia da comportamenti irresponsabili e condotte illegali che non possono essere validamente contrastate se mancano le risorse. I tagli al bilancio del Ministero e al sistema delle aree protette, fra le quali rientrano le aree marine protette che il disegno di legge n. 979 in esame intende responsabilizzare, sono patrimonio acquisito dei pareri parlamentari e preoccupano, per le ricadute concrete che essi determinano, i senatori di tutti gli schieramenti. Nella finanziaria 2009 proprio le aree marine protette hanno visto una contrazione di risorse per oltre 2,5 milioni di euro. Se qualcuno ha denunciato che per la prima volta negli ultimi dieci anni questa estate è trascorsa in più di un tratto di costa senza il servizio di pattugliamento, prevenzione e pronto intervento antinquinamento delle navi del Ministero dell'ambiente (anche perché la convenzione con il consorzio d'imprese che se ne occupa sembra sia stata rinnovata solo a fine luglio), la riduzione delle unità adibite a controllo rischia di vanificare le norme esistenti contro gli sversamenti in mare di idrocarburi, derivanti da incidenti o da atti dolosi come il lavaggio illegale delle cisterne, consolidando un rischio permanente per l'ecosistema marino-costiero ma anche e soprattutto per il turismo. Siamo quindi di fronte ad un problema che presenta una dimensione macro, (le attività criminali in senso stretto o gli sversamenti illegali delle grandi petroliere) ed una micro, cioè le conseguenze della pressione turistica e dell'affollamento delle imbarcazioni da diporto durante la stagione estiva, oppure le irregolarità

Si pensi che non sono operative molte aree protette, anche marine, la cui istituzione era stata progettata, ma non è attuabile per mancanza di fondi idonei (ce ne sono oltre una decina in questa situazione). Peraltro, il danno di immagine che il moltiplicarsi di fenomeni di inquinamento determina è sicuramente superiore, in termini di ricaduta sul turismo nazionale ed estero, al risparmio che si consegue nel singolo anno per le casse dello Stato. E se è assai dubbio che siano di giovamento nel contrastare i fenomeni di illegalità le recenti norme transattive volute dal Ministero dell'ambiente in materia di danno ambientale, è invece certo che che i progetti di riforma delle intercettazioni telefoniche aiuteranno, al converso, se approvati, le organizzazioni che dell'inquinamento hanno ormai fatto un *business* lucroso quanto carico di minacce per il futuro del patrimonio naturale italiano. È quindi un bene porre il problema di una eccessiva pressione turistica e antropica che alcuni tratti di costa, in particolare le isole minori, le aree marine protette e le aree marine di reperimento, sono costretti a subire durante il periodo estivo. La situazione infrastrutturale di tali aree, che pregiudica per certi versi anche una loro corretta gestione, sarà oggetto in Commissione lavori pubblici della riforma del settore portuale, che occorrerà monitorare con attenzione anche per le ricadute di attività quali la nautica da diporto o la balneazione. Nel frattempo occorre essere consapevoli della necessità di non varare nuove norme che abbiano un effetto diverso - non diciamo opposto, ma diverso - rispetto a quello desiderato. Se, come sembra, il disegno di legge mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera, che doti i tratti di costa sottoposti ad una pressione diportistica stagionale pericolosa per l'ecosistema (in particolare per il fondale marino, minacciato dagli ancoraggi indiscriminati) di campi di ormeggio attrezzati *off shore* per l'attracco, il rischio è che si determini una eterogeneità e difformità di situazioni tale per cui si avrebbe, da un lato, l'opzione per il divieto assoluto di ancoraggio e, dall'altro, un moltiplicarsi di campi boe a seconda della sensibilità del singolo Comune. Il disegno di legge, infatti, oltre alle aree marine protette, coinvolge anche, all'articolo 2 e al comma 8 dell'articolo 1, anche altri enti e Comuni. Si unirebbe, in questo caso, il massimo di intransigenza (con effetti non desiderabili rispetto ad una realtà economicamente importante quale l'attività diportistica) con il minimo coordinamento tra i Comuni che dovessero scegliere di utilizzare questo o quel criterio per istituire e gestire i campi ormeggi, con un effetto a macchia di leopardo che ci fa richiedere un impegno del Governo ad assicurare in ogni caso un coordinamento, a livello tecnico, delle soluzioni adottabili. Si possono cioè creare situazioni pericolose:

Ora, occorre riconoscere anche che il testo ha subìto nel corso del suoi *iter* alcuni miglioramenti apportati ad opera dello stesso relatore, che poi coincide col proponente e primo firmatario, in ossequio ai pareri espressi dalle Commissioni consultive. In particolare, in luogo di un obbligo generale posto in capo ai Comuni, l'articolo 1, comma 1, reca ora la disciplina di una "possibilità" concessa agli enti gestori delle aree marine protette di istituire, con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, campi attrezzati sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto. Quella che ancora manca è una garanzia che le soluzioni concrete individuate da ciascun ente o Comune siano effettivamente idonee a perseguire le finalità delineate dal disegno di legge nella riduzione del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili, nell'erogazione di un numero non illimitato di permessi di stazionamento e nella trasparenza di accesso. avvio a concludere, signora Presidente. In tale quadro non è neppure chiaro come i Comuni possano coerentemente operare sulle aree marine di reperimento, vale a dire le aree per le quali è in vista l'istituzione di una area protetta, data la natura ibrida dello *status* di questi territori. In alcuni casi la prospettiva di riscossione di una tariffa potrebbe, in assenza di coordinamento nazionale, portare anche a soluzioni ambientalmente non soddisfacenti, specialmente alla luce della pesante penalizzazione che i bilanci comunali hanno conosciuto negli ultimi anni. intervento dicendo che, rilevati gli aspetti di indeterminatezza del provvedimento in esame, pur dopo le modifiche apportate, si intende concludere che nessuna efficace ed efficiente tutela dell'ecosistema marino sarà possibile nella perdurante tendenza a ridurre gli stanziamenti a favore dell'ambiente (oggi scesi a meno dell'1,5 per cento delle risorse pubbliche destinate all'ultima manovra finanziaria) e nessuna area protetta, marina o terrestre, potrà garantire investimenti nello sviluppo di sistemi di salvaguardia innovativi finché le risorse statali ad essa dedicate serviranno, come nella situazione attuale, a coprire solo la spesa corrente, ammontando, nel loro complesso, a meno di due terzi del fabbisogno reale. Presidente, prima di svolgere qualche breve considerazione sul provvedimento di cui è primo firmatario il senatore Ranucci,

utili elementi di riflessione per orientarci anche sui lavori del Senato, su come dovremo proseguire la nostra attività nel corso della legislatura. Credo sia molto importante che nel Senato si dibattano grandi questioni politiche e che sia giusto anche affrontare le grandi riforme.

che le grandi questioni del Paese siano affrontate dal Parlamento. Credo anche che sia utile e che serva seguire l'attività legislativa del Governo Governo ed i modi in cui in Parlamento il Governo opera per attuare il proprio programma. Ma non credo, Presidente, che faccia bene al Senato ed al Parlamento che l'attività legislativa di iniziativa parlamentare venga trascurata come accade in Senato.

Non credo nemmeno che sia utile e che faccia bene ai lavori del Senato la trascuratezza con cui il Governo tratta la nostra attività ispettiva,

e non se ne accelera la discussione e la votazione. Non possiamo continuare a relegare a margine della nostra attività elementi costituzionalmente decisivi per il Parlamento;

mi conferma in questa opinione anche il contenuto dei provvedimenti di cui ci occupiamo in questo avvio di legislatura.

perché tende a dare una buona regolamentazione ad una parte di quel fenomeno turistico che oggi sta

di imbarcazioni, grandi e piccole, che con i loro ancoraggi stanno distruggendo la flora dei nostri fondali. Questa è una situazione gravissima,

al turismo di massa. Abbiamo bisogno del turismo di massa, siamo favorevoli allo sviluppo del turismo popolare ed al movimento delle persone e siamo molto favorevoli ai

In una grande città come Roma, con una struttura urbanistica in parte barocca, in parte rinascimentale, ricca di reperti le strade del centro storico, che sono adatte esclusivamente al traffico delle carrozze e dei cavalli, perché sono state costruite per questo, oggi vengono ingombrate quotidianamente

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che l'Aula si appresta a votare rappresenta, crediamo, un momento importante della politica italiana, poiché frutto di sereno confronto e positivo dialogo, condizioni che sempre dovrebbero caratterizzare i rapporti fra partiti seri e responsabili. Tale atteggiamento, comunque, si verifica già in seno alla Commissione ambiente, di cui mi onoro far parte, ove la propensione al dialogo è pratica ricorrente e costituisce esercizio naturale e poco faticoso, conseguenza diretta delle qualità umane e politiche dei miei colleghi, oltre che della sagacia, esperienza ed equilibrio di chi la presiede. Desidero, pertanto, ringraziare vivamente i colleghi dell'opposizione, senatore Raffaele Ranucci e senatore Roberto Della Seta,

Un esempio positivo di come si possa lavorare in sinergia superando steccati ideologici o di partito per affrontare e risolvere tematiche di interesse collettivo. Nel merito, il disegno di legge in esame ha la finalità di tutelare l'ecosistema nelle isole minori e nelle aree marine di pregio, di cui è ricco il nostro Paese, consentendo, nel contempo, a dette aree una oculata fruizione turistica da cui oggi sono escluse. Inoltre, prevedendo la possibilità di creare campi ormeggio in tali zone, il disegno di legge ha la fondata pretesa di costruire un nuovo modello di sviluppo economico ed occupazionale che ruota attorno al turismo. Infatti, nella logica che precedeva tale disegno di legge erano presenti poche aree di tutela, belle e pulite, ma quasi inaccessibili. Ed in tale logica di divieto, e dei parchi marini come sinora concepiti, si racchiudeva il concetto che «altrove si può fare» quello che non è consentito nei parchi. Col presente disegno di legge vengono, viceversa, individuati altri luoghi costieri da tutelare, ma da rendere fruibili in maniera oculata. Un principio, quindi, vantaggioso per l'ambiente, l'economia e l'occupazione. Sul testo elaborato dal senatore Ranucci sono stati apportati e condivisi emendamenti migliorativi che renderanno ancor più qualificante ed efficace il risultato. Particolarmente, si è tenuto conto del fatto che il nostro sistema paesaggistico, per quanto vasto, è tra i più delicati e, pertanto, un eccesso di pressione antropica e turistica potrebbe rischiare di comprometterne il valore. In tal senso, il disegno di legge, nel regolare i flussi, mira a dotare le isole minori e le aree marine di pregio di parchi boe ed ormeggi che consentiranno di tutelare il fondale marino, eliminando gli ancoraggi nelle praterie di posidonia, permettendo, oltre a ciò, una corretta fruizione del litorale, con la valorizzazione di posti e paesaggi prima sconosciuti. Per il turista, quindi, una prospettiva diversa di conoscenza del territorio, un angolo di osservazione complementare e la possibilità di scoprire ed ammirare i paesaggi proprio dal mare, favorendo la fruizione integrata parchi boe-ormeggi e territorio. Quanto sopra previsto non costituirà un obbligo per i Comuni, cui sarà devoluta, invece, la possibilità di istituire tali campi ormeggi. In ultimo, signora Presidente, siamo felici, pur non possedendo barche a vela, che il disegno di legge in esame abbia tenuto conto anche delle esigenze e dinamiche della nautica velista e del settore *charter*, avendo evitato che tali comparti potessero risultare penalizzati, pur rappresentando il turismo migliore e più rispettoso dell'ambiente. *(Applausi

intervengo per una brevissima replica. Volevo dire al senatore Di Nardo che siamo assolutamente d'accordo sul fatto che le risorse per

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 1.100, l'opportunità che, per i comuni, l'istituzione dei campi-ormeggi ivi previsti sia configurata come possibilità e non come obbligo». come possibilità e non come obbligo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo l'articolo 3 venga aggiunto il seguente: "Art. 3-*bis*. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Sugli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.109, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

a sottolineare una carenza dell'articolo. La legislazione vigente di natura costituzionale

associazioni private, che non possono assolutamente gestire il demanio marittimo turistico in regime di esenzione concessoria). Analizzando le aree marine protette istituite e affidate in gestione,

ad associazioni privatistiche, che sono associazioni naturalistiche di un certo spessore, come il WWF, ma sempre privatistiche rimangono:

mio voto contrario sull'emendamento 1.100 scaturisce dall'approfondimento che la Commissione ha fatto anche con l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e con i rappresentanti delle Capitanerie di porto. La questione che solleva il senatore De Angelis può essere sicuramente affrontata in futuro alla luce della possibilità

la Commissione si propone di affrontare - così come dirò nella dichiarazione di voto finale sul provvedimento - nel corso di una revisione della legge n. 394 del 1991, che presiede alla disciplina delle aree marine protette. non sono mai state sollevate eccezioni sul fatto che le aree marine protette, peraltro di assoluta competenza statale, anche alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, possano essere

vorrei che si individuasse esattamente il punto in cui inserire al comma 3 la competenza dei Comuni a dare l'intesa. Mi permetto di osservare

**Il Senato non approva.**

esaminato l'AS 979 recante istituzione di campi di ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine dimaggior pregio ambientale e paesaggistico; tenuto conto che uno degli obiettivi basilari del provvedimento è quello di tutelare le aree marine maggiormente sensibili e delicate

offerti alle attività turistiche; preso atto che la riqualificazione e lo sviluppo turistico dell'isola di Lampedusa sono arrestati, oltre che dai problemi di carattere sociale legati agli sbarchi degli extracomunitari, anche e soprattutto dalla carenza delle infrastrutture nautiche e da diporto e dalla mancanza di porti turistici attrezzati; impegna il Governo ad autorizzare un apposito contributo per l'isola di Lampedusa, anche a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, ai fini della realizzazione di un porto turistico, da realizzare in area da definire da parte delle autorità competenti anche attraverso le procedure di *project financing* di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Senatrice Maraventano, Presidente, con il Presidente della Commissione avevamo concordato l'impegno del Governo. Signora Presidente, il Presidente della Commissione non può assolutamente impegnare la volontà del Governo, ma solamente esprimere un'opinione in sede di dichiarazione di voto.

Nelle aree marine di reperimento i Comuni possono istituire campi di ormeggio con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509

è esploso a Kabul un mezzo militare italiano, e vi sono stati almeno tre morti nelle nostre Forze armate,

e soprattutto di chiedere al Ministro degli affari esteri e a quello della difesa di venire a riferire in Senato in tempi brevi, perché la gravità e la reiterazione dell'episodio meritano un adeguato approfondimento da parte del Parlamento.

già risposto alla mia richiesta. imprecise ma certamente drammatiche, che stanno giungendo. Si tratta di una missione che ha il compito di difendere i valori della libertà e della democrazia. Come tutti siamo in attesa

Colleghi, in attesa che il Governo venga a riferire, sospendo la seduta fino alle ore 11. La seduta è sospesa.

in un grave attentato terroristico. Il numero delle vittime e dei feriti non è stato ancora accertato in modo definitivo, ma purtroppo, dalle notizie ancora frammentarie finora pervenute, sembra ormai certo che ci siano almeno sei militari italiani morti e altrettanti feriti. Anche a nome del presidente Schifani, che, come sapete, assolve la funzione di supplente del Capo dello Stato, esprimo, certa di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, il più profondo cordoglio per le vittime dell'attentato,

La seduta è sospesa.

ho subito voluto, prima di ogni dichiarazione ai *media*, venire in Parlamento per riferire ai parlamentari e quindi al Paese

dove il nostro contingente opera con circa 450 militari. Con due mezzi «Lince», che più di una volta hanno salvato la vita ai nostri soldati, stavano percorrendo la strada che conduce dall'aeroporto alla città quando sono stati oggetto di un

hanno tutti subìto le conseguenze dello scoppio: sei hanno perso la vita e quattro sono rimasti feriti. Le prime notizie mi dicono che non versano in imminente pericolo di vita, ma tali notizie devono ancora essere confermate. Abbiamo naturalmente già i nomi di coloro che purtroppo hanno perso la vita, ma poiché le famiglie non sono state ancora tutte avvertite, mi consentirete che su questo mantenga il doveroso riserbo. Posso solo dirvi che hanno perso la vita quattro caporalmaggiori, un sergente maggiore e l'ufficiale, un tenente che comandava i due Lince. Le parole di cordoglio non sono mai in questi casi, specie per il Ministro della difesa, adeguate, ma sono sicuro di interpretare, veramente, il pensiero non solo di tutto il Governo, non solo delle alte gerarchie militari, ma di tutti gli italiani nell'esprimere la vicinanza vera e profonda alle famiglie dei caduti, ai loro comandanti e a tutti coloro che stanno operando in condizioni difficili in quello scenario internazionale dove i nostri soldati stanno facendo fino in fondo il loro dovere con orgoglio, con passione, con forte motivazione morale, anche a costo dell'estremo sacrificio della vita. Io recentemente sono stato a trovarli e sono rimasto veramente colpito dalla loro serenità, dal loro coraggio, dalla loro determinazione, dalla loro consapevolezza non solo del rischio che correvano e che corrono, ma anche dalla loro piena comprensione della missione che stanno svolgendo lontano dai confini della Patria non solo per la ricostruzione di quello sfortunato Paese, ma anche a tutela della nostra libertà contro il il terrorismo. Agli infami, vigliacchi aggressori che hanno colpito ancora una volta nella maniera più subdola sicuramente la nostra ferma convinzione che non ci fermeremo nelle valutazioni che con tutto il il consesso internazionale abbiamo fatto e continueremo a fare, mai isolatamente ma insieme agli organismi internazionali che questa missione hanno deciso e che vogliono continuare.

Signora Presidente, intervengo brevemente a nome del mio Gruppo e personalmente per partecipare al cordoglio e al grave lutto. Anche il nostro intervento e il nostro cordoglio non sono sicuramente formali. In momenti gravi come questi è importante l'unità del Paese per superare tutte le difficoltà. Chiediamo un'attenzione che non sia formale, rituale anche nei confronti delle famiglie.

in questa situazione anche a livello di Stato perché anche loro lunedì scorso hanno perso due persone. Il Governo aveva avuto qualche difficoltà a rapportarsi perché

si prova un grosso senso di disagio. Intendo, come il Ministro, fare un ragionamento serio. La situazione è delicata; facciamo in modo di agire unitariamente; cerchiamo di ragionare con serenità su quello che bisogna fare.

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, una giornata iniziata con il sole si è spenta di prima mattina con le notizie che arrivano e che lei, signor Ministro, ci ha confermato. Ringrazio il Governo per aver accolto l'unanime invito a riferire a botta calda, quindi con un sussulto di sentimenti e di passioni che ci coinvolgono, perché quanto è accaduto ci colpisce e ci induce peraltro a ragionare insieme. opportuno che, dopo questa comunicazione, come quella analoga che ella, signor Ministro, farà nel pomeriggio all'altro ramo del Parlamento, il Parlamento tutto venga coinvolto in un dibattito su questa particolare missione che l'Italia sta svolgendo in quella parte del mondo. Noi preannunciamo in proposito una mozione perché il Parlamento discuta e discuta subito. Non si tratta solo di rifinanziare le missioni. Noi siamo stati favorevoli a farlo perché sapevamo che i nostri militari avrebbero dovuto continuare a partecipare ad una missione che per noi doveva rimanere di pace, con tutte le garanzie e con tutta la sicurezza possibili. Ma oggi non basta. Dobbiamo approfondire e capire se esistano ancora le ragioni per una nostra permanenza. è una polemica in un momento particolare; è la volontà di stimolare in tutti noi, a partire da chi vi parla, una riflessione dura. Vedete, è nelle cose la riflessione. Ormai le elezioni in Afghanistan si sono svolte e la stessa Unione europea

per essere fedeli a quanto dice la nostra Costituzione, dobbiamo essere con le nostre straordinarie

ad un dittatore se ne sostituisca un altro e la lotta non sia più tra la democrazia e la dittatura, ma tra il dittatore e i talebani. Non è questa la funzione che l'Italia deve svolgere. in una missione di pace, dare sostegno a quelle popolazioni. Il signor Ministro, il Governo, noi tutti, sappiamo che le missioni di pace si fanno in maniera diversa, dando supporti formativi, supporti sanitari, supporti industriali. Si tratta di un'altra forma di presenza. È questa che noi dobbiamo valutare; questo dovrà valutare il Parlamento in una seduta apposita da prevedere. I minuti di silenzio non possono essere così frequenti. I minuti di silenzio ci richiamano ad un sussulto di ragionevolezza. La nostra intelligenza sa che i nostri uomini non possono essere sacrificati. Abbiamo nei confronti dei nostri soldati la massima stima.

i familiari delle vittime e coinvolge tutti noi. Diamo buona, grande e sincera testimonianza se ragioneremo delle vite di coloro i quali ancora sono nei posti difficili in cui il Parlamento li ha mandati,

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto partecipare il dolore profondo del mio Gruppo e mio personale per l'evento tragico di oggi in cui hanno perso la vita rappresentanti delle nostre Forze armate in Afghanistan. Forse la prima domanda a questo punto da rivolgere, con la ricerca di una rassicurazione, al ministro

alcune proposte e domande al ministro La Russa, al Governo e alla maggioranza. È ovvio che la questione riguardante la nostra presenza in Afghanistan - come dice il ministro La Russa è concordata costantemente con gli organismi internazionali. Non è polemico dire che un grande Paese, di fronte a questa responsabilità, ha la necessità e il dovere di trovare una maggiore forza in una relazione continua, anche nel dibattito parlamentare, con le opposizioni. con le opposizioni. Ho sentito i toni di questo piccolissimo dibattito e ho visto anche una dichiarazione del Presidente della Commissione difesa della Camera, rappresentante della Lega. Credo che dovremmo approfittare della riflessione e del dolore a cui ci conduce l'evento di oggi per svolgere una discussione in Parlamento meno rapsodica di quanto non accada sulle missioni internazionali e su quella dell'Afghanistan; meno rapsodica e - mi permetto di dire - anche alla presenza del Ministro degli affari esteri. Molti fatti politici sono maturati in questo mese: il più evidente, quello che abbiamo dinanzi agli occhi, sono le elezioni; le contestazioni dell'Unione europea; la conferenza stampa del presidente Karzai e, qualche ora dopo, l'attentato che ha colpito le nostre Forze armate; di un mese e mezzo fa che i Governi di Germania, Gran Bretagna e Francia hanno indirizzato al Segretario generale dell'ONU con la quale hanno chiesto una conferenza internazionale da svolgersi entro l'anno proprio sull'Afghanistan.

la nostra presenza negli organismi internazionali e le nostre determinazioni, ma soprattutto offrono all'Italia uno spazio politico di rilievo internazionale per poter su questi percorsi di decisione interferire e veramente codecidere. La morte di sei persone è sempre un fatto che appare deserto, infecondo; lo spegnimento di una vita è, in sé, la cessazione della fecondità. Proprio però, Proprio però, la responsabilità di fronte a queste morti, a questi ferimenti e anche, lasciatemelo dire, al rischio e alla paura (sentimento assolutamente umano, che va sempre insieme al coraggio, perché sia coraggio vero)

alla nostra azione che riguarda le missioni internazionali di pace e l'Afghanistan, sia sotto il versante delle politiche affidate al ministro La Russa

che valgano non solo all'Italia il ruolo e la gratitudine internazionale che le spettano, anche per il sacrificio che sta compiendo in Afghanistan, ma anche un ruolo, una forza e una capacità di codecisione negli organismi internazionali, che talvolta ci è apparsa appannata.

onorevoli senatori, è il momento del dolore e del cordoglio, che certamente non ci esime da riflessioni sulla politica. Come Gruppo del Popolo della Libertà esprimere la nostra partecipazione sofferta, sbigottita, addolorata a questo nuovo lutto delle Forze armate, uno degli eventi (se anche il numero delle

ai caduti di Nassiriya. In quella occasione (era la ricorrenza di quel terribile attentato), i volti dei loro familiari, dei loro figli ci mostrarono ancora una volta, nelle sale del Senato, il dolore e la sofferenza, che resta indelebile anche ad anni di distanza,

Ci rattrista pensare ad altri volti e ad altre famiglie che in queste ore sono raggiunte da telefonate e comunicazioni così drammatiche.

tutti gli elementi per le riflessioni che alcuni hanno abbozzato e che svilupperemo ulteriormente. Vogliamo, in primo luogo, stringerci intorno alle Forze armate, alla Folgore, che da quello che si dice è il reparto colpito, così carico di storia, di sofferenze, di eroismi.

quelli che oggi sono caduti e quelli che sono impegnati in tante parti del mondo. Chi li ha conosciuti, chi ha visitato questi reparti, i vari Governi che si sono succeduti e che in tante occasione sono stati accanto, vede come essi siano convinti di quello che fanno ed anche come i riconoscimenti ai militari italiani non riguardino solo il piano militare della sicurezza ma anche il piano umanitario, del soccorso alle popolazioni, ai bambini, alle famiglie, soprattutto - potrei dire - in Afghanistan, dove questa missione dura da anni e dove i riconoscimenti sono stati tanti. Crediamo quindi (ma ne discuteremo nelle occasioni che doverosamente il Parlamento, il Governo e la comunità internazionale dovranno dedicare a tali eventi) che dobbiamo difendere le ragioni di quei ragazzi, di quei militari e di quei reparti, donne e uomini, che sono impegnati in Afghanistan e altrove e che lo fanno con grande fierezza ed orgoglio, sapendo di servire una causa giusta. Conosciamo gli scenari politici dell'Afghanistan: non è forse questo il momento e l'occasione, almeno così riteniamo, per analisi dettagliate sulle elezioni, sui dibattiti e su tutti i messaggi oscuri ed inquietanti che il terrorismo fondamentalista invia, con una cronologia precisa, seguendo le vicende elettorali e politiche.

una funzione importante. Le ragioni della libertà e le ragioni della democrazia sono quelle per cui quel popolo ha votato giorni fa e non sono dalla parte di chi, con le autobombe, va a stroncare le vite dei militari. Difendere le ragioni della libertà e della democrazia è una cosa giusta, anche se costa un prezzo: è sempre stato così nella storia. Discuteremo, chiederemo l'allargamento di questo dibattito nella sede internazionale, un coinvolgimento di altri Paesi. La libertà e la democrazia in Afghanistan e in altre parti del mondo non sono questioni che riguardano la Folgore, il Governo italiano e la nostra Nazione riguardano la comunità internazionale. Oggi lasciateci piangere con quelle famiglie. Ci sarà poi il tempo della politica. Oggi è il tempo del dolore e dell'abbraccio alle nostre Forze armate.